L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, ricorre oggi l'anniversario della strage di via dei Georgofili. Questa mattina ho ricevuto la signora Giovanna Magiani Chelli, portavoce dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage. A lei, certo di aver interpretato in tal modo il sentimento di tutta l'Assemblea, ho espresso la solidarietà commossa del Senato, insieme con l'impegno a far sì che vengano reperite le risorse finanziarie necessarie ad assicurare un pronto ed adeguato risarcimento del danno alle vittime dei reati di tipo mafioso. Anche così ritengo si può contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. **Sul

festeggiamo oggi i cinquant'anni di attività parlamentare del nostro autorevole e stimato collega Francesco Cossiga, che nel 1958 - III legislatura - divenne deputato e dal 1983 senatore della Repubblica. La sua storia politica, iniziata già nel 1944 quando aderì alla Democrazia Cristiana, si caratterizza, come a tutti noto, per due elementi fondamentali: l'aver ricoperto, nessuno escluso - unico tra i politici italiani - i più prestigiosi incarichi di governo ed istituzionali, fino alla Presidenza del Senato e quindi all'elezione a Capo dello Stato; e l'essere stato tra i più giovani della storia repubblicana ad assumere la responsabilità di questi alti uffici. In ogni fase della sua intensa attività pubblica, il legame con la propria terra e la propria gente, con la sua Sardegna, è stato un elemento di orgoglio, di riconoscimento ideale e di identità. Un legame così profondo che ha rappresentato per la stessa terra sarda un motivo di vanto ed ulteriore, preziosa conferma della ricchezza della sua storia, della antica bellezza della sua lingua, della sua letteratura, della sua tradizione giuridica e culturale. Di quello spirito alto, fiero e nobile, il senatore Cossiga è stato interprete fedele ed appassionato testimone in Italia e nel mondo. Nel rivolgergli, a nome di tutta l'Assemblea, e mio personale, il più cordiale augurio per la felice ricorrenza, desidero al di là di ogni ulteriore nota biografica ricordare come nelle diverse circostanze che hanno segnato il suo impegno civile siano stati il «primato della politica» ed il «primato della coscienza» gli assi portanti della sua presenza nelle istituzioni. Già in uno scritto del 1951 il senatore Cossiga - che di lì a poco avrebbe visto riconosciuto dalla comunità accademica il valore scientifico dei suoi studi - con chiarezza e lucidità preveggenti riconosceva nella «effettiva partecipazione della base popolare alla vita dello Stato il supporto e l'anima» della democrazia. Nelle approfondite e densissime "Note sulla libertà d'espatrio e d'emigrazione" del 1953, considerava «ogni limitazione alla libertà personale» l'espressione di un rapporto tra «un interesse dell'ordinamento e 1'interesse dell'individuo». Il primato della politica era per lui, oggi come allora, l'espressione più alta di una tensione etica dell'agire civile al quale dovevano informarsi tanto i rappresentanti del popolo sovrano quanto gli stessi cittadini. Quel primato rappresenta il vincolo di reciprocità più forte tra eletto ed elettore, garanzia di tenuta dell'intero sistema di relazioni democratiche e civili. Per il politico, però, il primato della coscienza rappresentava un qualcosa di più e per molti aspetti irrinunciabile: il pungolo ed il monito a non arretrare mai di fronte alla coerenza dei valori e dei principi condivisi. Il primato della coscienza è la costante di uomini ai quali il senatore Cossiga si è sempre dichiarato idealmente debitore: Tommaso Moro e il suo compagno di prigione John Fisher, il cardinale John Henry Newman, Antonio Rosmini, solo per citarne alcuni. La libertà di coscienza nella sua riflessione e presenza parlamentare non è mai apparsa una scorciatoia imboccata per eludere i problemi nella loro immediata incidenza storica, bensì il criterio di giudizio - severo e rigoroso - di ogni scelta e di ogni iniziativa. Sembrano perfettamente consonanti le parole di quello che, a ragione, il teologo Bruno Forte addita come "l'avvocato della coscienza", Alfonso de Liguori: «la libertà è il requisito necessario della moralità». Una libertà indissolubilmente intrecciata con il senso di responsabilità verso gli uomini e verso il proprio Paese. Libertà e responsabilità da viversi nella testimonianza diretta e quotidiana, da non relegarsi a formule vuote solo dichiarate e non coerentemente realizzate. Davvero nelle parole dei suoi interventi in Aula, che tutti noi colleghi abbiamo potuto ascoltare, e dove egli contribuisce nei momenti più significativi ad arricchire il dibattito politico, si percepisce quel senso del dovere etico e civile che rimane ancora oggi pratica concreta e vera di amore per le istituzioni. La sincerità delle sue parole affiora in modo esemplare, a tratti commossi, quando il suo pensiero si rivolge ai nostri militari impegnati in missioni di pace all'estero. A loro si rivolge chiamandoli "nostri ragazzi" e loro, dalla sua voce e dalla sua tenace, fedele difesa, si sono sentiti sempre "figli della Patria", orgoglio di tutti noi e dell'Italia intera. Grazie senatore Cossiga. Tanti cari e affettuosi auguri, Presidente!

Signor Presidente, le sono grato per aver voluto che il Senato ricordasse che, il 26 maggio 1958, io entrai per la prima volta a far parte del Parlamento nazionale, essendo stato eletto alla Camera dei deputati per la circoscrizione della Sardegna, nelle liste della Democrazia Cristiana, cui ero già iscritto dall'età di 16 anni; e la ringrazio anche per le parole che ha voluto rivolgermi. E così, in quell'ormai lontano giorno, entrai in un Parlamento nel quale dal Regno di Sardegna, al Regno d'Italia e poi alla Repubblica italiana, mi avevano preceduto altri sardi: il barone Giuseppe Manno, presidente del primo Senato di Torino, noto anche per aver votato scendendo dallo scanno perché temeva che la mozione a favore della politica estera di Cavour fosse bocciata; il reverendo Giovanni Spano, il reverendo Giorgio Asproni, radicale e repubblicano; Pasquale Umana, Francesco Cocco-Ortu, Emilio Lussu, Antonio Segni, Bobore Mannironi e Antonio Maxia. Un Parlamento che, da erede del Parlamento di Torino, molto deve, per la Costituzione e un regime rappresentativo, ai rivoluzionari sardo-piemontesi, tra i quali mi onoro di avere un mio avo, eroe del Risorgimento, don Efisio Tola, tenente della Brigata Cremona di stanza a Chambery, una delle tre capitali del piccolo Regno, fatto fucilare, per ordine di re Carlo Felice di Savoia, sugli spalti di quel castello insieme a granatieri, fanti e carabinieri, poi gettati in una fossa comune dal cui anonimato furono tratti per l'amore che nutriva per l'Italia un grande Presidente della Repubblica francese, François Mitterand, che nel cimitero di quella città fece erigere sulla fossa comune un monumento dedicato ai martiri e anche apporre una nobile targa in ricordo del mio antico prozio. Mi trovai perciò, indegnamente, a sedere alla Camera dei deputati, insieme agli amici e maestri Giulio Andreotti e Aldo Moro, già personaggi eminenti, prima che nel nostro partito e nel Parlamento, nella FUCI, il movimento degli universitari cattolici italiani, di cui furono presidenti, che tanta parte ha avuto nella formazione culturale e politica della classe dirigente, politica ed amministrativa della gloriosa Prima Repubblica. Nel 1983 fui eletto senatore ed entrai così a far parte di questo ramo del Parlamento dove non votai mai, perché fui eletto tosto Presidente del Senato. Vi fu poi il settennale intermezzo della Presidenza della Repubblica, per me e per il Paese infausto e senza frutti, perché flagellato da una campagna di disprezzo, di calunnie e di denigrazioni, una sorta di *damnatio memoriae* in vita, condotta da uomini politici ed in particolare dalla stampa di un potente gruppo editoriale italiano sotto la guida di un presuntuoso voltagabbana (dal fascismo al razzismo e dal monarchismo al socialismo) e perciò squallido. Costui fu non amato «compagno di strada» del di lui ben più nobile Partito comunista italiano, ma, a dire il vero, non come invece lo fu il suo padrone, «compagno di strada» - per interesse materiale - non solo del Partito comunista italiano, ma anche dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e del KGB. Parentesi infausta - dicevo - perché, per la prima volta, un Presidente della Repubblica fu offeso e vilipeso con epiteti ingiuriosi da cortei di massa, senza che mai la magistratura intervenisse, e per ben due volte si tentò di trascinarlo davanti alla Corte costituzionale in sede penale e dovette giustificare il suo operato davanti a Commissioni d'inchiesta e, cessato dalla carica, fu anche processato dal Tribunale dei ministri. Con un senso di liberazione lasciai il Quirinale e, in data 28 aprile 1992, rientrai a far parte del Parlamento nazionale, la mia casa, in questo Senato, anche se solo in forza di una che considero anacronistica disposizione costituzionale. Ebbi l'onore di collaborare con Giovanni Leone, Mariano Rumor, Carlo Donat-Cattin; con Amintore Fanfani, Paolo Emilio Taviani, Benigno Zaccagnini e Ciriaco De Mita, *leader* preminenti di quel grande partito di popolo che fu la Democrazia Cristiana, la cui storia di servizio al Paese e alla democrazia è consegnata allo storia e non può certo essere infangata da qualche magistratuncolo - come si tentò di fare - o da qualche registucolo, inopinatamente premiato da chi può essere anche nostra consorella, ma certo non benevola amica: la Nazione latina d'oltralpe. Fu per me un onore sedere in Parlamento accanto a Palmiro Togliatti, il grande *leader* politico del «partito nuovo», che studiò, tra l'altro, nel mio stesso liceo, abitò lungamente nella mia città e - guarda caso

preservò l'Italia da una guerra civile devastante, dopo che il nostro Paese aveva combattuto contro i tedeschi invasori quella grande guerra patriottica che fu la Resistenza, anche fermando quella guerra civile e di classe che, in nome di una irreale visione della posizione dell'Italia, di tante vittime fu causa, non solo ex appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana, ma anche antifascisti, partigiani, militari del Regno del Sud, preti seminaristi, ragazzi del movimento cattolico, che furono uccisi in nome di un'utopia che poi, in nome di una Resistenza tradita ed incompiuta,

accanto a Pietro Nenni, a Giuseppe Saragat, a Randolfo Pacciardi, a Ugo La Malfa e Oronzo Reale, a Giovanni Malagodi e anche a Giorgio Almirante, cui l'Italia molto deve perché, attraverso la parlamentarizzazione dei giovani di Salò, come li chiamò giustamente l'amico Violante, avviò il processo di inserimento nella democrazia coloro che erano stati fascisti o militanti nella Repubblica di Salò. Tale processo fu iniziato a sinistra grazie alla larga (e di grande respiro) amnistia concessa da Palmiro Togliatti, guardasigilli dell'epoca, contestato duramente dal suo stesso partito, per i reati commessi durante la Resistenza da partigiani, ma anche da membri delle Forze armate della Repubblica Sociale Italiana. Ciò che poi portò all'adesione di massa di ex militari della Repubblica Sociale Italiana al Partito comunista italiano in numeri che superano, come scrissero gli storici comunisti, 36.000 appartenenti. E voglio ricordare che ebbi l'onore di sedere accanto ai rappresentanti delle minoranze nazionali: da Severino Craveri, grande *leader* valdostano, a Toni Ebner, a Roland Ritz e a Karl Mitterdorfer, asso della Luftwaffe, difensore di Düsseldorf da attacchi aerei terroristici - ahimè! - da parte degli Alleati, tedeschi del Tirolo del Sud, che con la loro prudenza e saggezza contribuirono a collocare la loro Nazione, parte culturalmente della grande Nazione germanica e storicamente della Nazione austro-tedesca, accanto a quella italiana, di lingua francese e slovena, nel quadro unitario e democratico della Repubblica italiana. E fu per me un onore immenso far parte di queste Camere del Parlamento nazionale, di quel sovrano legale da cui ogni legittimo potere civile, militare, giudiziario deriva, come affermò in un grande discorso Palmiro Togliatti nell'Aula della Costituente, quando prese la parola per opporsi a che l'ordine giudiziario fosse chiamato potere giudiziario, affermando che potere non poteva essere perché emanava da un concorso e non dalla sovranità popolare. Ché quando il fascismo volle spazzare via la democrazia rappresentativa e il regime di libertà spazzò via il Parlamento con le leggi del 1926 ed i partiti, non le Forze armate, non la Polizia e neanche la magistratura, che di fatto aderì nella quasi totalità al regime, mandando in galera Pajetta, Terracini, De Gasperi, Lussu, Amendola e tanti altri ancora. Perché mai nella storia né giudici né Corti costituzionali, dall'Austria alla Repubblica di Weimar, furono di ostacolo all'avvento delle dittature - giammai! - cui si opposero o tentarono di opporsi, invece, solo i liberi Parlamenti. La generazione della Prima Repubblica, che non ha lasciato eredi, se non qualcuno nel Partito Democratico, nell'Unione di Centro e in Alleanza Nazionale, ha passato la mano ad una nuova generazione: quella dei Berlusconi, dei Bossi, dei Veltroni, dei Fini e dei Di Pietro. Non siedono più in Parlamento i grandi partiti popolari: la Democrazia Cristiana, il Partito comunista italiano e il Partito socialista italiano che, insieme ad antichi partiti democratici quali il Partito repubblicano e il Partito liberale, insieme all'allora piccolo ma, come già dissi, di grande utilità per lo stabilimento di un regime democratico partecipato da tutti gli italiani, il Movimento Sociale Italiano, radicarono la democrazia e il regime delle libertà nel nostro Paese. Certo - e non è falsa modestia, perché chi mi conosce sa che modesto certo non sono, anzi piuttosto presuntuoso, almeno intellettualmente - non grande è stato il mio contributo alla vita e alla storia del Parlamento e delle istituzioni repubblicane, anche perché io non godevo e non godo certo dell'autorità intellettuale di un Einaudi o di un Segni o di un Leone, di un prestigio politico quale quello di Gronchi, di Saragat e di Pertini o dell'altissima autorevolezza e prestigio morale di Scalfaro e di Ciampi, ed oggi con una fortunata sintesi goduto dal presidente e mio collega Giorgio Napolitano. Sono passati i tempi in cui Giorgio Napolitano ed io apparimmo in televisione, in una trasmissione intitolata «La politica dei giovani»; quando incontro Giorgio Napolitano non abbiamo il coraggio di riguardare la cassetta. Molte le accuse che mi sono state rivolte, come quella di aver concorso a costituire bande armate. Certo, sono stato giudicato dal Tribunale dei ministri per formazione di banda armata e attentato alla sicurezza dello Stato, reati per cui in tempo di guerra è prevista la pena di morte con fucilazione alle spalle. Sono stato accusato di essere stato un favoreggiatore di terroristi per solidarietà con un compagno di partito e, infine, tesi avvalorata dall'attuale Ministro dell'interno, di aver complottato con i *commandos* della Marina militare, cui appartengo da ufficiale di complemento a titolo onorifico. Mai, neanche dall'avventuriero fascismo giudiziario, fui accusato di essere un ladro o un malversatore o comunque uno che ha approfittato delle numerose, anche se solo quasi per caso, cariche ricoperte. Quello che posso dire è che sono entrato al Palazzo del Viminale più ricco di quanto ne sia uscito; sono entrato a Palazzo Chigi più ricco di quanto ne sia uscito; sono entrato al Quirinale più ricco di quanto ne sia uscito. E ho collaborato a falcidiare le mie proprietà, dopo che già erano state colpite dalla riforma agraria, votando a favore, con un appassionato discorso, della riforma dei contratti agrari. Ricordo che la mia grande povera sorella, che non c'è più, quando la sera andai a cena da lei mi fece trovare sotto il tovagliolo, che come in tutte le case le case del Meridione e delle Isole stava sul tavolo, il conto esatto di quanto io le avevo fatto perdere. Sono certo che, abbattuta la Prima gloriosa Repubblica per grandi fatti epocali la cui origine costituisce ancora un quasi mistero, terminato senza successo il tentativo di instaurare una Seconda Repubblica, Repubblica, con sagge ed appropriate riforme, nel quadro dei principi fondamentali della Costituzione del 1948, questo Senato e il Parlamento intero riusciranno ad instaurare la Terza Repubblica. Questo è il mio augurio.

Signor Presidente, a nome mio e del Gruppo che ho l'onore di presiedere, anche grazie al presidente Cossiga, voglio associarmi alle sue parole nei confronti di un uomo che con la sua attività politica, parlamentare ed istituzionale rappresenta una parte importante della nostra vita repubblicana. Credo di poter dire che per tantissime italiane e italiani il presidente Cossiga è un esempio e le sue opinioni, anche quando non condivise o scomode, stimolano in profondità il dibattito giuridico, politico e culturale del nostro Paese. Per noi giovani, poi, rappresenta un modello di impegno politico ed istituzionale e ci consegna quotidianamente una semplice ed importante lezione: mai fermarsi alla superficie delle cose, leggere i fatti sempre, anche quando sono scomodi, e avere il coraggio di dire ciò che si pensa. Per noi democristiani, poi, il presidente Cossiga è un particolare motivo di orgoglio, anche per quel sottile gusto dell'invettiva, che ci è mancato in passato e che forse, insieme ad una maggiore dose di coraggio, ci avrebbe consentito di cambiare un po' il corso della nostra storia. Un ringraziamento particolare, signor Presidente, da parte dei colleghi sudtirolesi e valdostani per le parole di apprezzamento e di stima e per il lavoro al servizio delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche che lei ha svolto e svolge nella sua attività parlamentare. Se mi è consentito, un ringraziamento personale anche per aver scoperto in queste settimane un antico legame di consuetudine familiare che mi rende ancor più felice di farle oggi a nome del Gruppo e mio personale tanti auguri per la sua attività parlamentare, che ci auguriamo sia ancora più lunga di quella che lei non abbia già svolto.

mezzo secolo di vita parlamentare per il presidente emerito, senatore Francesco Cossiga, e che vita, è il caso di dire, ripensando alla sua irripetibile biografia, che ha attraversato i fenomeni ed i momenti più alti e più drammatici della metà del secolo scorso: lo ha ricordato molto bene nell'intervento il Presidente emerito. Tracciare il profilo del senatore Cossiga è compito arduo, specie se in poche parole si avesse la presunzione di richiamare i mille salienti episodi che lo hanno visto protagonista: dagli incarichi di Governo più prestigiosi, sino alla Presidenza del Consiglio ed al Quirinale, del quale è stato un degnissimo, anche se discusso, inquilino. Ma forse, anche per la memoria di questi giorni, vale la pena di ricordare il suo dramma umano e politico consumato con il rapimento e l'assassinio del presidente della Democrazia Cristiana - il suo partito - Aldo Moro. Spesso, con disperata commozione, il senatore Cossiga ricorda quei giorni nei quali i sentimenti umani più nobili furono costretti a fare i conti con la ragion di Stato. Ma ricordiamo soprattutto, chi come me e come tanti di noi è di un'altra generazione, il suo modo unico di interpretare il ruolo del politico a tutto campo; campo; uno dei pochi della cosiddetta Prima Repubblica che, dall'alto dello scranno del Quirinale, ha cominciato a capire che questo sistema non funzionava più così come era stato concepito. Il suo modo pronto a staffilare chiunque, amico o avversario che fosse, e pronto anche a cambiare opinioni, come capita a chi ha avuto in dono un'intelligenza di primo ordine. Siamo certi che il contributo del senatore Cossiga continuerà ad essere di sicura qualità, di altrettanta chiarezza ed autenticità, perché Francesco Cossiga insegna a tutti noi cosa significa essere uomini liberi e voi sapete quanto la libertà di espressione sia cara al nostro movimento. *Ad* *multos* *annos*, senatore.

Signor presidente Schifani, la sua decisione di celebrare i cinquant'anni di impegno parlamentare del senatore Cossiga ha un rilievo particolare: segna un omaggio doveroso della nostra Assemblea ad uno dei suoi componenti più illustri, ma offre anche a tutti noi la possibilità di svolgere qualche considerazione, che troverebbe altrimenti difficile ospitalità nei nostri dibattiti. al presidente Cossiga il sentimento molto particolare con il quale molti di noi ascoltano i suoi interventi. Ammiriamo la sua cultura, la precisione straordinaria con cui ricorda la nostra storia (ne abbiamo avuto un esempio poco fa), la lucidità della sua analisi politica, l'efficacia laser e la tempestività con cui riesce a definire il suo pensiero. Conosciamo anche il suo spirito democratico e la sua lealtà verso le istituzioni repubblicane; ma c'è di più. Molti di noi nascondono un'invidia positiva, un'invidia rivelatrice, per la libertà e l'indipendenza con la quale il presidente Cossiga manifesta le sue posizioni politiche, mai cedendo alla retorica o a quella genericità verso la quale noi, purtroppo, tanto spesso, per calcolata prudenza o per vizio di conformismo, rischiamo di scivolare. Il presidente Cossiga ha deciso di privilegiare la verità e ci ha abituati a sentirgli dire quello che pensa: quello che pensa: per questo suo stile dobbiamo ringraziarlo particolarmente, perché ci ricorda che nessun Paese può andare lontano se i suoi leader non esprimono le loro posizioni in modo franco e leale. Agli auguri dei senatori del Partito Democratico voglio aggiungere i miei auguri personali, e spero che i colleghi senatori mi consentiranno di farlo, perché risale agli inizi degli anni Settanta la mia prima collaborazione con Francesco Cossiga, allora ministro per la riforma della pubblica amministrazione; una collaborazione poi proseguita al Ministero dell'interno e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Cossiga ha dato prova di possedere sia la necessaria sensibilità politica sia quelle doti di uomo di Stato e di uomo dello Stato senza le quali mai dovrebbe essere possibile governare le istituzioni. Adesso, dopo quasi trent'anni nei quali, sempre per scelta democratica del Parlamento, il presidente Cossiga, cattolico liberale, ha rivestito le più alte cariche della nostra Repubblica, è per me motivo di grande onore poter sedere con lui nei banchi del Senato. Ma ricordare i cinquant'anni della sua vita parlamentare, così lunga e tanto ricca ed interessante, mi porta ad una riflessione di carattere più generale - non me ne voglia, Presidente su questa nostra Italia che da troppo tempo si è come rassegnata a trascurare quei cittadini che più hanno vissuto e quindi più possono dare, che non investe più né sugli anziani né sui giovani. È così che il Paese va verso il declino: signori senatori, non aiutare i giovani nelle cui mani è riposto il nostro avvenire, altrettanto grave è non sentire il bisogno di valorizzare adeguatamente quel patrimonio di conoscenze, di esperienze, di equilibrio, di saggezza, di cui è portatore chi non è più giovane. L'esempio del presidente Cossiga, la qualità e lo straordinario rilievo del suo apporto intellettuale alla vita politica e culturale del nostro Paese, ci ricordano che abbiamo il dovere di restituire a tutti i cittadini che non sono più giovani quel ruolo sociale e culturale cui hanno diritto e di cui noi abbiamo un grandissimo bisogno. Auguri carissimi, presidente Cossiga.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor presidente Cossiga, a nome del Gruppo del Popolo della Libertà mi associo ai voti augurali che tutti le rivolgono oggi in quest'Aula, sottolineando il ruolo prezioso e fondamentale che lei ha svolto nella ormai lunga ma ancora aperta al futuro esperienza politica da protagonista di primo piano. Del resto, le sue parole, i riferimenti, le citazioni, gli intrecci

e i 50 anni di impegno in politica dimostrano che, in un'epoca ormai non vicinissima, lei è stato un esponente di nuove generazioni che all'età di 30 anni si accingevano a dare un contributo importante alla vita politica e istituzionale. Oggi, mentre si parla molto della necessità di un rinnovamento generazionale, ciò dimostra che in epoche ormai non vicine nuove generazioni ebbero la possibilità di cimentarsi e di essere in prima linea nell'azione politica.

al '68, in quel '77 che fu anno di grandi sconvolgimenti nella vita italiana seppe assumersi responsabilità difficili, a volte non comprese, molte volte criticate da destra o da sinistra, ma che - rilette a trent'anni di distanza - diedero un contributo importante alla difesa della legalità repubblicana e dell'ordine nella nostra Nazione. Voglio anche ricordare il Cossiga ministro dell'interno che nel 1978 - domani si ricorderà in quest'Aula Aldo Moro

esperienza politica - con un gesto che ebbe un valore simbolico, in qualche modo sottolineò la drammaticità di quei momenti più volte ricordati in questi giorni in cui ricorre il trentennale dell'eccidio di Moro e della sua scorta. Tutti ricordiamo il senso dello Stato, la sofferenza con cui il presidente Cossiga affrontò quel momento drammatico della vita italiana. Ricordiamo poi Cossiga presidente del Senato. Ricordiamo Cossiga - lo ha detto lui stesso, e lo ringrazio personalmente - come l'uomo del dialogo che, a sinistra come a destra, diede un contributo essenziale al processo di legittimazione democratica che oggi possiamo dire definitivamente compiuto e che deve molto all'opera del politico Cossiga che ringrazio sentitamente per le parole che pronunciò, per gli atteggiamenti che assunse,

Credo che questa sia stata un po' una civetteria per farsi dire pubblicamente che in quegli anni e soprattutto nella parte finale del suo mandato il suo coraggio nel parlare, il suo "piccone" diedero un contributo importante all'avvio di una stagione di rinnovamento. un altro difficile momento di passaggio della vita repubblicana, con le sue parole, il suo "piccone", il suo spirito iconoclasta, che ogni giorno faceva sobbalzare nei palazzi della politica e nelle redazioni dei giornali i parlamentari, i ministri, i giornalisti pronti a smontare le prime pagine dei quotidiani per dare il giusto risalto alle sue affermazioni forti e vigorose, forti e vigorose, lei, avvertendo l'incedere dei tempi, ha dato un contributo essenziale al rinnovamento della politica che noi ci auguriamo, proprio in questa legislatura, con un bipolarismo maturo, sappia vivere un momento importante di antagonismo democratico, ma di civiltà del confronto alla quale lei ha fatto sempre riferimento. In queste vesti molteplici voglio ringraziarla per alcune citazioni e alcuni riferimenti. Lei ha ricordato il suo rapporto con Giorgio Almirante, di cui quest'anno ricorre il ventennale della morte. In una fase non facile della vita politica lei seppe sempre coltivare la civiltà del dialogo dialogo e del rispetto, aprendo la strada ad una stagione di democrazia più matura e avanzata. La ringraziamo anche per questo e anche per ciò che di tanto in tanto leggiamo sui giornali,

che ha pronunciato come protagonista della storia, ma anche come uomo che all'interno delle istituzioni ha saputo vedere sia le cose buone sia quelle che negli anni hanno avvelenato la vita politica italiana e non sempre sono state superate. Quante vicende! Ne ricordo solo una, perché mi è rimasta vivida nella memoria: quell'agosto del 1980 - ero consigliere regionale - in piazza, a Bologna, dopo la strage della stazione,

che commettono le stragi e gli omicidi, ma soprattutto con coloro che, stando al Governo e cercando di contrastarli, si vedono addossate responsabilità che non sono loro. Quante responsabilità sono sono state addossate e quante ce ne ha ricordate il senatore Cossiga! Eppure le cose che ha detto sono assolutamente sagge e condivisibili: una su tutte, la centralità del Parlamento, che raramente viene ricordata in questo Paese, come sede della sovranità popolare e unico luogo nel quale davvero si esprime la democrazia. Parlamento troppe volte aggredito storicamente da altri poteri o da altri ordini (chiamiamoli come vogliamo), che anche oggi - ahimè, basta sfogliare i giornali - viene

sicuramente è stato notato da tutti, dall'estrema sinistra all'estrema destra; quante lotte, quanti contrasti veri, quante visioni diverse in politica estera, quante visioni della società diametralmente opposte, ma quanta civiltà in Parlamento, da Togliatti ad Almirante, ai *leader* repubblicani, liberali, socialisti, democratici cristiani, nel rispetto reciproco, sia pure nella diversità delle posizioni. È stata una piccola lezione di storia e di saggezza: spero, presidente Cossiga, che, oltre agli applausi di tutti i senatori immagino - anche di tutti i deputati, ci sia anche la convinzione di seguirla in alcune delle indicazioni che ci ha dato per il passato e che vanno trasferite nel futuro.

ovviamente che questi apparecchi vengano custoditi e restituiti all'elettore dopo il voto e che, per chiunque contravvenga a questo divieto, l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 300 a 1.000 euro. Evidentemente la norma è dettata dall'allarme suscitato nell'imminenza delle elezioni, dalla possibilità che alcuni elettori usino questi strumenti per rendere non più segreto il loro voto e di conseguenza per fare degli usi certamente proibiti dalla legge e in particolare dalla Costituzione, come, ad esempio, praticare la vendita di voti o subire un'imposizione da parte di qualcuno che con la forza, con minacce, con lusinghe, con pagamenti possa richiedere a qualcun altro di votare in un certo modo e di portargliene la prova. [**Presidenza sia prima sia dopo le elezioni, di casi in cui questo è effettivamente avvenuto (per la verità si è parlato di casi avvenuti prima delle scorse elezioni) e pertanto è stato certamente un atto un atto opportuno da parte del Governo Prodi l'aver emanato questo decreto. La data del decreto stesso, il 1° aprile e cioè a meno di due settimane dalle elezioni, testimonia essa stessa l'urgenza. Quanto alla necessità, è evidente. Giustamente, la premessa al decreto-legge cita, accanto agli articoli 77 e 87 della Costituzione (quelli che disciplinano il decreto-legge e i poteri del Capo dello Stato per quanto riguarda la sua autorizzazione a presentare tale forma di norme), anche il secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione, che per l'appunto prescrive che il voto debba essere personale ed eguale, libero e segreto. Se viene meno la segretezza del voto, tendono a venir meno anche le altre tre caratteristiche dettate dalla Costituzione: infatti, se il voto non è segreto può non essere più libero e se non è libero di fatto non è più personale, non è più nella disponibilità del singolo elettore, che può trovarsi costretto a cedere, sostanzialmente, la possibilità di votare, attraverso un voto obbligato e controllato, ad altre persone, il cui voto finisce per non essere eguale a quello degli altri, perché ne controllano un numero maggiore. Vorrei aggiungere ancora un aspetto dal punto di vista costituzionale. È evidente che un decreto-legge in materia elettorale non potrebbe essere emanato se riguardasse i meccanismi attraverso i quali i voti vengono trasformati in seggi o in maggioranze o in elezione di singoli candidati: in questo caso si tratta di un aspetto per un verso organizzativo e per un altro di tutela di uno dei requisiti essenziali del voto finalizzato ad una emergenza che si è venuta a creare, o meglio che è venuta ad essere percepita, nell'imminenza delle elezioni. Un altro aspetto che val la pena ricordare è che questa norma, che forse sarebbe stato meglio introdurre nell'ambito del Testo unico per le elezioni della Camera dei deputati - che costituisce sostanzialmente un testo base per tutte le elezioni le elezioni per le norme che non riguardano i singoli aspetti delle elezioni di altri livelli - è stata formulata come a sé stante proprio perché riguarda tutte le elezioni, incluso il referendum, e dunque anche le elezioni regionali che, sulla base della nuova formulazione approvata nel 1999 dell'articolo 122 della Costituzione, dovrebbero essere competenza regionale. Trattasi però di un aspetto di carattere generale, della tutela di un aspetto costituzionale particolarmente delicato e fondamentale per la garanzia di tutte le altre elezioni che il Governo ha ritenuto essere nelle proprie competenze, citando espressamente la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e cioè la competenza statale sulle norme di carattere penale. Un'ultima considerazione in ordine all'efficacia di questo provvedimento: certamente è stato efficace; ha rappresentato certamente un forte deterrente nei confronti di coloro che

maggiori indagini sulla presenza di questi strumenti, che ormai possono essere molto piccoli e possono essere usati di conseguenza in cabina con una certa facilità.

dovrà studiare un sistema per ridurre ulteriormente la possibilità di violare il segreto del voto;

anche se la materia andrà riesaminata allo scopo di rendere lo sforzo di tutela della segretezza del voto pienamente efficace. finestra"). Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

le disposizioni attinenti alla segretezza del voto. È evidente, signor Presidente, colleghi, che esso contiene in se tutti i presupposti della necessità e dell'urgenza.

e che pertanto si richiami espressamente ai presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Il provvedimento in esame interviene su un fenomeno che, come abbiamo potuto constatare, negli ultimi anni

eguale, libero e segreto. Questa previsione costituzionale era sicuramente esposta a violazione dato dato che, molto spesso, non solo le cronache giornalistiche ma anche moltissime indagini giudiziarie ci hanno mostrato come ci siano stati fenomeni di condizionamento del voto

di associazioni criminali e malavitose e si sono registrati, appunto, fenomeni di voto di scambio non solo acclarati dalle cronache giornalistiche, ma anche da molte indagini giudiziarie.

ci informasse sull'entità materiale del fenomeno: sappiamo che c'è stato, ma non ne conosciamo la configurazione. Potrebbe essere utile sapere quanto è stato vasto e come è stato colpito, fondamentalmente per tenere sotto controllo il processo che determina il fenomeno del voto di scambio.

I mezzi elettronici privati possono rappresentare un mezzo di controllo del voto di scambio, ma il voto elettronico rischia di tradursi in un metodo di falsificazione sistematica del voto. Quindi,

Si è sempre ritenuto che in materia elettorale in senso stretto, per ciò che attiene dunque la formula elettorale e il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, non si possa procedere attraverso lo

si dà il via libera ad un decreto-legge, che non riguarda la formula elettorale - lo ripeto, materia inibita - ma la legislazione elettorale di contorno e dunque tutto ciò che non è strettamente legato alla trasformazione dei voti in seggi. Il fatto che non si sia nell'ambito della formula elettorale ma della legislazione elettorale di contorno, non vuol dire però che si sia in un ambito irrilevante o secondario rispetto alla formula elettorale. Infatti, come sostiene il professor Enrico Grosso, nel più recente commento all'articolo 48 della Costituzione, la legislazione elettorale di contorno è costituzionalmente obbligatoria e di particolare rilievo complessivo per il rispetto dei princìpi dell'ordinamento. dell'ordinamento. Il secondo punto è stato già in parte accennato dal collega Malan. I quattro aggettivi con i quali l'articolo 48 della Costituzione definisce il voto si richiamano a vicenda: personale ed uguale, libero e segreto. Vanno quindi interpretati in modo circolare. La segretezza è la prima garanzia per la libertà del voto, libertà dal controllo sociale anche al di là della volontà specifica dell'elettore. Infatti, nella nostra legislazione elettorale di contorno sono cinque le garanzie principali: la previsione di una scheda di Stato, che lo Stato quindi stampa secondo determinate caratteristiche (articolo 31 del Testo unico della Camera dei deputati); la previsione di una cabina elettorale dove votare segretamente (articolo 58 la punizione del presidente del seggio o di chiunque impedisca l'ingresso dell'elettore nella cabina (articolo 111); il divieto di voto palese o l'esibizione della scheda o di segni di riconoscimento (articoli 58, 62 e 70); il numero

che non vanno mai diminuite, ma vanno sempre preservate e, caso mai, aggiornate. Il terzo punto è rappresentato dall'applicabilità a tutte le consultazioni.

stabilisce che in materia elettorale le Regioni hanno competenza, ma nell'ambito dei princìpi stabiliti con legge dello Stato. Di conseguenza, in questo caso siamo in presenza di una normativa che rientra a pieno titolo perché è applicazione diretta dell'articolo 48 della Costituzione; del resto, l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), stabilisce che in materia penale l'intervento dello Stato è esclusivo. quarto ed ultimo punto, vorrei non dimenticassimo anche un altro aspetto già accennato dal collega Malan. Mi riferisco al fatto che altre parti della segretezza del voto vanno tutelate in altre normative e pongono problemi *de iure condendo*. primo è quello già segnalato rispetto al voto all'estero. Nel voto all'estero la segretezza del voto è garantita oggettivamente, ma non soggettivamente

sulla spedizione dei plichi elettorali (sia che li riceva effettivamente colui che ha diritto di voto, sia che siano spediti effettivamente da colui che ha diritto di voto) e in terzo luogo anche sulle procedure di spoglio vanno ulteriormente precisati. precisati. Un altro punto delicato sulla segretezza del voto è quello relativo al referendum, di cui all'articolo 75 della Costituzione. Infatti, l'utilizzazione tattico-strategica dell'astensionismo,

Quindi, andare a votare in cabina elettorale non è di per sé una garanzia di segretezza proprio per questo motivo. Pertanto, va rimeditata la questione del *quorum*. Il *quorum* attuale, costruito al 50 per cento più uno degli aventi diritto, è stato pensato per una situazione in cui votava

funzionamento anche per i limiti alla segretezza del voto. Pertanto, nell'ambito del ripensamento sulle garanzie dello statuto dell'opposizione, anche l'abbassamento del *quorum* a soglie più ragionevoli, come la metà più uno dei votanti alle precedenti elezioni politiche, è materia di cui tutti noi dovremmo preoccuparci.

praticato anche da noi - attraverso il quale al mattino un elettore si impadronisce di una scheda autentica sostituendola con una contraffatta, anche malamente, e la

sistemi usati. Sappiamo che il nostro Paese è tra i migliori per quanto riguarda la tutela della regolarità delle elezioni. In ogni caso, è necessaria una costante vigilanza. Raccolgo anche l'osservazione del senatore Pardi sul voto elettronico. Credo che l'espressione ed il conteggio dei voti attraverso un procedimento elettronico siano molto rischiosi. Ricordo una proposta fatta nella scorsa legislatura dall'allora

qualcuno renda riconoscibile il proprio voto, anche quando non si deve esprimere una preferenza, dove ci si può sbizzarrire nei segni di riconoscimento, e dove è necessario apporre solo un segno per indicare il partito che si intende votare, agli elettori un timbro che lascia sempre lo stesso segno. Di conseguenza è assolutamente irriconoscibile un voto rispetto ad un altro. Ringrazio, infine, il senatore Ceccanti per il suo approfondimento di carattere costituzionalistico e generale sulla questione della segretezza del voto, sulla quale credo davvero dovremo ritornare per una tutela maggiormente stringente.

Presidente, tutti quei provvedimenti che migliorano ed aumentano - come in questo caso - le condizioni e le garanzie sulla segretezza del voto sono da salutare favorevolmente anche perché in essi vi è un richiamo ad un rigore istituzionale. In una stagione nella quale l'antipolitica cavalca ogni occasione e ogni pretesto, è bene che il Parlamento e, in particolare, il Senato della Repubblica, offrano un'immagine di democrazia piena e di trasparenza. A ciò si aggiunga che l'impegno non deve limitarsi al presente provvedimento, ma deve avviare una politica che sappia garantire il funzionamento delle Camere.

se riusciamo a sommare questo nuovo rigore con la novità di un Ministero per la semplificazione legislativa, allora il Parlamento potrà essere visto non solo come il luogo più alto della democrazia rappresentativa, ma anche come una preziosa fucina capace di porsi in sintonia con i cittadini.

all'interno di un quadro di regole e di norme che devono ispirarsi sempre ai princìpi e ai valori della democrazia rappresentativa. Pertanto, il voto del Gruppo Lega Nord Padania al

Signora Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del Partito Democratico voteranno a favore del

anche nella mia città, a Catania, casi in cui elettori ricevevano un anticipo di 50 euro e la consegna di un telefonino, con il quale entravano nella cabina elettorale

deterrente nei confronti di un fenomeno di malcostume che è molto grave e che non conosce latitudini. Per queste ragioni i senatori del Partito Democratico voteranno a favore. Anche noi auspichiamo, ancora una volta, che siano votati altri e più incisivi strumenti che consentano di tutelare la segretezza del voto e nello stesso tempo di impedire fenomeni di compravendita dei voti, ahimè assai diffusi nel nostro Paese, in particolare in alcune Regioni. *(Applausi

viene introdotto il reato elettorale attraverso l'uso del telefonino. Sono materie legate all'innovazione tecnologica. Certamente dieci anni fa non si sarebbe pensato ad un provvedimento di questo genere. Bisognerà capire come la tecnologia potrà influire, anche in futuro, sul sistema elettorale e soprattutto sull'espressione del voto.

una congrua distinzione, facendo presente che non si può intervenire con decreto-legge quando si va a stabilire una relazione fra il voto e il seggio ma riconoscendo che i dettagli organizzativi possono essere affidati ad uno strumento di urgenza.

da scegliere per evidenti ragioni di necessità. Credo che la discussione su questo provvedimento, sia alla Camera che al Senato, sia stata utile.

i due rami del Parlamento, è stata posta in essere una discussione che, come dicevo all'inizio, si è dimostrata estremamente interessante.

Presidente, mi rendo conto che quello che dico ha uno scarsissimo interesse, quindi da parte mia chiedo perdono ai colleghi senatori, tuttavia la ringrazio per il suo cortese e garbato intervento. Come stavo dicendo, in questa legislatura ci

tanto più in quest'Aula del Senato ci fa ben sperare per tutto quello che potremo realizzare nei prossimi cinque anni, che io mi auguro estremamente fecondi. Ribadisco pertanto il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà.

Presidente, colleghi e rappresentanti del Governo, soltanto oggi pomeriggio abbiamo potuto sviluppare

un approfondimento adeguato sui temi del trasporto pubblico locale, che sicuramente sono rinviati ad altri momenti, perché meritano tutta l'attenzione dovuta. Malgrado questo, in occasione di

Il disegno di legge consente di erogare un contributo di 80 milioni di euro alla società Trenitalia spa, interamente di proprietà del Tesoro,

della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale

fa parte dell'erogazione alle Regioni per il successivo riparto, anche se è subordinata all'effettuazione successiva dello stesso. Siamo in presenza di una materia estremamente complessa, che è in questo momento subordinata a trasformazioni anche molto recenti, quali la direttiva comunitaria emessa il 30 aprile 2008 in ordine alla regolazione della aiuti di Stato alle società di trasporto ferroviario. Essa è poi soggetta a tutto il processo di liberalizzazione del trasporto passeggeri, che non è ancora avviato (mentre, come sapete tutti, è stato avviato il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario delle merci).

per una serie di rapporti contrattuali inerenti al trasporto ferroviario. L'ultima finanziaria consente infatti alle Regioni di ricavare dalle accise sui carburanti le risorse necessarie per affrontare questo tema, ma esse sono esentate fino al 2010 dall'intrattenere un rapporto con Trenitalia. In questo quadro si colloca il decreto, che quindi determina un aumento di 80 milioni di euro, o meglio, una quota di 80 milioni di euro all'interno degli incrementi rispetto alle risorse stabilite sin dal 2000 a

impostato un ampio dibattito in Commissione ed è intervenuto il parere favorevole della 1a Commissione permanente. Questo è il tema di cui oggi dobbiamo discutere. Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che i tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi. È iscritta a parlare la senatrice Incostante per 16 minuti. Ne Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, come ha ricordato il relatore, autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'anno di esercizio 2008 per garantire, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto ferroviario regionale in concessione a Trenitalia. La somma stanziata è corrisposta direttamente a quest'ultima società. Sul provvedimento, quindi, niente da eccepire, se non per quanto attiene l'indeterminatezza dei fabbisogni effettivi e per gli standard da onorare con i contratti di servizio e, soprattutto, circa la copertura temporale del fabbisogno per l'anno in corso. Nel provvedimento, infatti, si parla dei primi mesi del 2008, senza definire con precisione la scadenza temporale oltre la quale l'erogazione dei servizi non risulta coperta e sarà pertanto necessario intervenire con un ulteriore provvedimento. Va da sé che ritengo personalmente deplorevole porre a raffronto la situazione ereditata nella scorsa legislatura con quella attuale, dove altri furono i termini delle consegne ricevute ed altri i problemi cui porre soluzione. di nuova fase si deve trattare (gli eventi poi ci diranno per quanto), sarebbe auspicabile che il nostro sguardo fosse rivolto al futuro e si volgesse indietro solo per prenderne riferimenti utili e non certo per attizzare il fuocherello della polemica sterile e fine a se stessa, che già tanta distanza a mio avviso ha prodotto tra i cittadini ed i loro legittimi rappresentanti. Proprio per questo, signor Presidente, avevamo chiesto in Commissione uno slittamento della trattazione del provvedimento nella giornata di domani, per poter approfondire questioni non irrilevanti circa la natura e la durata della copertura di servizi che hanno un grande impatto per la collettività e per i nostri concittadini, quali quelli dei trasporti ferroviari regionali, che interessano ogni giorno (è bene ricordarlo) oltre 15 milioni di nostri concittadini. Come ho premesso in Commissione, non vi era da parte nostra nessuna pregiudiziale (non ci poteva essere) sul provvedimento, né intendevamo esaurire l'intera complessità della materia, come ricordava appunto il relatore, con un provvedimento ordinario come il disegno di legge di

infatti, costituisce non soltanto un'apprezzabile inversione di tendenza nel passaggio di consegne tra due Governi a cavallo della legislatura, ma anche un tassello di un processo di riforma complessivo. di una riforma strutturale del trasporto pubblico locale che data ormai da oltre un decennio e che nel nostro Paese, nonostante l'alternarsi di diverse maggioranze, non si è mai completata; mi auguro pertanto che questa sia l'occasione perché a partire dal provvedimento in esame si possa cominciare a ragionare attentamente sulla convenienza della conclusione di un processo di riforma che è iniziato negli anni Novanta e che non si è ancora concluso. Un percorso, lo ricordiamo, che ha preso le mosse dalla legge di riforma, con il decreto legislativo n. 422 del 1997. Fu infatti con tale provvedimento che venne disciplinato il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Le funzioni delegate alle Regioni riguardano, infatti, l'intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di interesse regionale e locale, e le competenze conferite sono essenzialmente di carattere programmatorio, amministrativo e finanziario. La Regione, dunque, è individuata come unico soggetto regolatore di tutto il comparto e ad essa è attribuita una doppia responsabilità, pianificatoria e finanziaria. In ossequio al principio di sussidiarietà le Regioni sono peraltro tenute a conferire a Province, Comuni ed enti locali in genere le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale. L'ultima legge finanziaria ha riformato ulteriormente il finanziamento del trasporto pubblico locale sostituendo il sistema di trasferimenti erariali alle Regioni con l'attribuzione alle stesse di risorse proprie derivanti da quote di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione erogato in ciascuna Regione. La finanziaria per il 2008, attribuendo autonomia finanziaria alle Regioni a statuto ordinario in relazione al finanziamento del trasporto pubblico locale, completa per così dire la riforma Bassanini del 1997. Non voglio, sia chiaro, magnificare gesta o tessere lodi improprie, ma solo confermare e rivendicare un modello coerente di riforma che ci ha guidato con coerenza in questi anni e su cui chiediamo e chiederemo, nelle settimane e nei mesi a venire, la possibilità di un confronto di merito per sfidarci reciprocamente, nel soddisfacimento del superiore interesse dell'utente cittadino ma non ancora cliente di questi servizi. Segnalo inoltre che la legge finanziaria per il 2008 stanzia 104 milioni per il contratto di servizio con Trenitalia per viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza e per i treni notturni. La legge finanziaria si occupa praticamente di tutto il sistema. Ad esempio, il comma 295 dell'articolo 1 riconosce alle Regioni a Statuto ordinario - come ricordavo - la compartecipazione al gettito dell'accisa del gasolio per autotrazione. Resta deficitaria soprattutto l'attenzione che è necessario rivolgere ai treni locali, in particolare quelli predisposti per i pendolari. Ricordo solo il comma 309 dell'articolo 1 della stessa legge finanziaria che reca una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore

Mi auguro però che vi sia anche un'unica politica che rimetta al centro i diritti di coloro che fino ad oggi sono considerati la cenerentola del trasporto pubblico in Italia: il trasporto locale e quello regionale, soprattutto su ferro. Nelle Commissioni parlamentari di competenza avremo sicuramente l'occasione di ascoltare le dichiarazioni programmatiche del ministro Matteoli. Lo attendiamo con impazienza e con curiosità perché siamo mossi dalla volontà di capire i suoi propositi anche su queste materie, per adesso molto latitanti rispetto a suoi pronunciamenti roboanti circa TAV, ponte sullo Stretto e grandi opere. Per intanto ci limitiamo ad esprimere doverosamente parere favorevole ad un provvedimento che consenta la parziale copertura dei servizi essenziali che - non dimentichiamolo (voglio sottolinearlo nuovamente) - ogni giorno consentono il trasporto di circa 15 milioni di cittadini che con essi si recano al lavoro o nei luoghi di studio e che spesso, purtroppo - come sappiamo non lo fanno in condizioni soddisfacenti in termini di pulizia degli ambienti, di orario di arrivo a destinazione e, più in generale, di comfort: scompartimenti troppo spesso freddi d'inverno e caldi d'estate. Un'Italia che vuole davvero essere un Paese moderno ed efficiente non può tollerare che si perpetui una condizione di servizio inaccettabile per la posizione a cui il nostro Paese vuole legittimamente aspirare.

*(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, siamo chiamati ad approvare queste disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali. È già stato ricordato che i pendolari, i cittadini, gli studenti che si svegliano la mattina presto, alle quattro e mezza, e che prendono i treni non sempre ricevono un servizio di qualità e all'altezza della situazione. Noi ci limitiamo semplicemente a verificare, per esempio, il monitoraggio di alcune associazioni dei pendolari e da tali verifiche constatiamo che i ritardi e le soppressioni dei treni sono molto consistenti. Ricordo, per esempio, che, solo su alcune tratte, l'anno scorso, nel

4.077 minuti di ritardo; a marzo, quattro treni soppressi e 4.186 minuti di ritardo: 13.308 minuti di ritardo in tutto. Bisogna dare servizi di qualità

come ho ricordato per quelli dei pendolari. Va chiarito quanta parte del fabbisogno 2008 il finanziamento aggiuntivo di 80 milioni, previa certezza dell'avvenuto versamento sul fondo di 96 milioni, previsto dal «milleproroghe», valga a soddisfare, atteso che nella relazione di accompagnamento si fa testualmente riferimento ai soli primi mesi di quest'anno. Occorre soprattutto chiarire in che modo sia possibile reintegrare quei capitoli da cui si prelevano le risorse indicate.

di Trenitalia un intervento di legislatura, che parta anzitutto dall'esigenza di individuare il perimetro di quel servizio universale che oggi è insoddisfacente

Signor Presidente, onorevoli senatori, a me preme mettere in evidenza un aspetto. Il decreto-legge, portando la data dell'8 aprile, cioè a soli cinque giorni dal voto, è inquadrato in una logica elettorale. Mi sembra doveroso metterlo in evidenza, perché i contributi alle

a contributi statali da erogarsi e aspettano. Questo saltare le procedure e avere atteggiamenti che non sono corretti mi sembra doveroso metterlo in evidenza, richiamando

per carità di patria e consapevoli anche del disagio e della necessità dei servizi, dobbiamo esprimere il nostro voto favorevole, con questo richiamando anche l'attenzione di chi ha proposto a suo tempo il decreto sul fatto che un conto è parlare di

un neoeletto mi sarebbe piaciuto approfondire ancor più la materia in oggetto. Ma ho ascoltato molto volentieri l'intervento del collega Filippi,

Per tali servizi le Regioni sono subentrate allo Stato nel rapporto con Ferrovie spa e hanno stipulato i relativi contratti di servizio. della legge n. 244 del 2007 (in sostanza la finanziaria 2008), è stata introdotta una riforma strutturale del sistema di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, che prevede la soppressione dei trasferimenti statali destinati al settore e la contestuale attribuzione alle Regioni di una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. In particolare, il comma 302 ha disposto che negli anni che vanno dal 2008 al 2010 continuino ad essere corrisposte le risorse destinate al finanziamento delle funzioni di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari regionali e locali in concessione a Trenitalia, trasferiti alle Regioni ai sensi del predetto articolo 9 del La norma che stiamo esaminando prevede una spesa di 80 milioni di euro per il 2008, da corrispondere direttamente alla società Trenitalia per garantire la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto regionale nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio e della rideterminazione dei criteri di ripartizione.

il territorio, le periferie si interrogano e ci guardano: questo è uno di quei momenti. Il servizio di trasporto locale è fatto male;

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui ci stiamo occupando riguarda un problema molto sentito soprattutto da parte delle persone che, quotidianamente, usufruiscono del trasporto ferroviario per spostamenti necessari per il lavoro, lo studio e le esigenze fondamentali di relazioni, di cura, di assistenza, e a garanzia del diritto a muoversi nel proprio territorio. Il trasporto ferroviario locale, non è una novità per nessuno, è un pò la parte più trascurata perché l'uso quotidiano ed intenso dell'automobile lo ha reso nel tempo meno visibile e di minore interesse. Ce ne accorgiamo solo quando i pendolari, esasperati, bloccano i binari e protestano con energia per la sporcizia, la mancata puntualità e le condizioni di sovraffollamento insopportabili con le quali devono fare i conti per poter svolgere il proprio lavoro e accudire la propria famiglia. Con questo provvedimento si assegnano a Trenitalia 80 milioni per la prosecuzione del servizio per il 2008. Si tratta di un provvedimento di natura transitoria e, per comprenderne bene l'esiguità e il carattere di assoluta emergenza, va inquadrato nella necessità di riprendere quanto prima un'attenta definizione delle risorse necessarie per un servizio ferroviario regionale all'altezza dei bisogni del nostro Paese e che risponda all'attesa di qualità dei cittadini. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento fa esplicito riferimento al completamento dei lavori del tavolo interministeriale a tal fine costituito e al successivo confronto con le Regioni, per quantificare, ripartire e garantire tempestivamente le risorse necessarie a mantenere il servizio. Per dare un'idea dell'ordine di risorse che servono per l'anno 2008, Trenitalia quantifica in 435 milioni di euro per i servizi di trasporto regionali contrattualizzati con le singole Regioni a Statuto ordinario. Nel 2007 queste risorse ammontarono a 334 milioni. Come si può ben vedere, 80 milioni servono solo per due o tre mesi. E il resto? Quando verrà erogato alle Regioni per poter continuare a fornire il servizio? Se si fa riferimento poi all'ammodernamento del materiale rotabile per il trasporto regionale, Trenitalia ha chiesto 230 milioni e non è stato reso disponibile nulla.

Il sottosegretario Castelli, nei giorni scorsi, ha sottolineato che le tariffe che pagano gli utenti sono troppo basse e che, se si vorranno servizi efficienti e di qualità, bisognerà prima di tutto mettere mano al portafoglio con conseguenti rincari che si riverseranno soprattutto sulle famiglie. Ricordo che stiamo parlando di servizi di trasporto che riguardano la pendolarità quotidiana per ragioni di lavoro e che coloro i quali li utilizzano hanno redditi medio-bassi, non in grado di sopportare rincari come quelli ipotizzati. La finanziaria del Governo Prodi ha introdotto la possibilità di detrarre il costo dell'abbonamento del trasporto locale dal proprio reddito imponibile; dico questo per mostrare quanto tale costo incida rispetto ad un reddito che è per sua natura molto basso. È opportuno quindi che il Governo chiarisca entro quale strategia intende utilizzare gli 80 milioni e se questi, come era nelle intenzioni del provvedimento, saranno il volano per il miglioramento ed il potenziamento del trasporto regionale ferroviario, nell'interesse di milioni di utenti e pendolari che hanno il dritto di poter viaggiare e muoversi utilizzando servizi degni di un Paese civile. Queste non sono preoccupazioni infondate e lo dimostra il fatto che, ad esempio, 1 miliardo e 400 milioni di euro per l'abbattimento dell'ICI sono stati distolti dal piano delle infrastrutture della Calabria e della Sicilia. È opportuno quindi che si faccia chiarezza sulla politica dei trasporti e delle infrastrutture di cui si intende dotare il nostro Paese. Ci auguriamo che i chiarimenti del Governo siano tempestivi

allontanare, almeno per il momento, il rischio di possibili ridimensionamenti dell'offerta del servizio ferroviario regionale e locale. Mi sia però consentito di ribadire qualche numero:

il conferimento alle Regioni di una sostanziale autonomia finanziaria nell'ambito del trasporto ferroviario regionale, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione,

alle Regioni della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione quale sistema per il finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale in previsione della stipula di contratti di servizio, il Governo Prodi non è riuscito a realizzare una sostanziale autonomia finanziaria, rinviando di fatto la questione al 2011, vale a dire all'entrata in vigore della riforma.

al sistema di finanziamento dei servizi ferroviari regionali e locali di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, affinché si possa arrivare, nel più breve tempo possibile, alla stipula dei nuovi contratti di servizio tra Regioni e Trenitalia

ascoltato con interesse le proposte ed il dibattito sul tema dei trasporti pubblici locali, vuole evidenziare il fatto che il decreto-legge in esame ha carattere di urgenza e riguarda un finanziamento particolare. Ritiene che

ma vuole porre l'attenzione sul fatto che si tratta di un decreto di finanziamento volto ad affrontare una situazione particolare di emergenza.

in previsione del fatto che dal 2011 tali servizi verranno finanziati secondo le quote di compartecipazione di ciascuna Regione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha infatti riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione quale sistema di finanziamento dei suddetti servizi.

a copertura degli oneri di servizio pubblico, mentre dall'anno 2011 tali risorse dovranno essere adeguate alle quote della compartecipazione al gettito dell'accisa, da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Se è vero, pertanto, che tale fonte di finanziamento conferirà una sostanziale autonomia finanziaria alle Regioni in materia, è pur vero che la precedente maggioranza di Governo ha scelto di seguire ancora per diversi anni la strada dei finanziamenti statali, rinviando l'entrata in vigore della riforma soltanto al 2011. In ogni caso, il nostro Gruppo esprime una posizione favorevole sul provvedimento ritenendo che, pur trattandosi di un finanziamento diretto a favore di Trenitalia spa, la misura possa per il momento allontanare il forte rischio di un ridimensionamento dell'offerta del servizio ferroviario regionale utilizzato dai nostri pendolari. Come dicevo prima, sono circa 2 milioni i pendolari che sopportano quotidianamente i gravi disagi legati ad un servizio ferroviario che ormai ha raggiunto veramente livelli di scarsissima qualità ed efficienza. È proprio di qualche giorno fa la notizia che la Corte dei conti, riferendosi al biennio 2005-2006, abbia constatato un sensibile peggioramento della qualità del servizio offerto dalla società Trenitalia in termini di pulizia, puntualità e disponibilità, nonostante il continuo incremento dei costi. Questo fatto è stato sottolineato anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. Alla luce di tali considerazioni si auspica, quindi, che la riforma introdotta con la legge finanziaria del 2008 possa trovare quanto prima compimento, riconoscendo alle Regioni una sostanziale autonomia finanziaria in materia; tale da poter restituire efficienza e competitività al trasporto ferroviario regionale e locale in favore degli utenti del servizio stesso

Presidente, colleghi, come già annunciato nell'intervento svolto in discussione generale, il nostro Gruppo non farà mancare il proprio voto favorevole al provvedimento in esame, che riteniamo assolutamente naturale da questo punto di vista. Voglio però richiamare l'attenzione dell'Aula, del relatore e del Presidente sul fatto che, nonostante il provvedimento abbia un carattere

mi hanno preceduto hanno ricordato l'importanza del servizio che riguarda ogni giorno oltre 15 milioni di cittadini su questo tema la nostra attenzione, la nostra vigilanza sarà ovviamente la più alta e la più intransigente possibile. Aspettiamo l'intervento del Ministro nella Commissione competente per capirne e valutarne

perché ci siamo convinti di votare a favore di tutti i decreti-legge presentati per farli diventare definitivamente legge del nostro Paese.

Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, una interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ieri il Consiglio comunale di Palermo ha negato l'approvazione di una delibera - che è stata ritirata oggi dal sindaco di Palermo - che prevedeva il raddoppio dell'addizionale IRPEF per il Comune di Palermo, in conseguenza della scelta del Consiglio dei Ministri, tenutosi a Napoli, di eliminare l'ICI.

destinate dal Governo Prodi per realizzare, per esempio, le metropolitane di Palermo, Catania e Messina, il secondo lotto della Agrigento-Caltanissetta; il nuovo attracco per il porto di Messina; il passante ferroviario di Palermo, opera quest'ultima che dovrebbe collegare i comuni dell'area metropolitana di Palermo, che si svilupperebbe per 30 chilometri, anche in sotterranea, con 8 stazioni, 18 fermate con un costo di 1.110 milioni di euro e con una previsione di conclusione lavori nel 2012.